Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per comprendere effettivamente come si intenda procedere con l'esame del disegno di legge sulla riforma della professione forense.

un interesse ad alcune modifiche del testo e alla riproposizione di alcuni emendamenti. Non è possibile che il dibattito parlamentare in Aula si svolga così stancamente e in modo asfittico. Vorremmo prima avere cognizione delle proposte che il relatore intende avanzare, e rispetto a queste iniziare un confronto serio, visto che quello fatto in Commissione evidentemente non è bastato, e non basta neppure tutto quello che è stato fatto fino a questo momento. con l'esame del provvedimento come tappabuchi per mettere un pezzo di professione forense su cui si continua a discutere e non si va mai avanti, quando ben altri sono gli intenti del relatore e del Governo,

nel nostro dibattito parlamentare che mi sembra senz'altro importante, visto che si deve rimediare a qualcosa che evidentemente è mancato

insieme al Governo e al relatore per capire se oggi sia necessario fare questa seduta, in che termini la vogliamo fare, o se ci sia bisogno invece di altro tempo per presentare

dimentichiamo anche il contenuto del precedente dibattito; siamo costretti a rimettere in discussione una serie di cose e davvero non mi sembra una maniera logica, corretta e ragionevole Quindi, chiedo subito che il relatore voglia darci le sue comunicazioni al riguardo. Mi appello al Governo perché a sua volta esprima il suo parere sul punto,

Noi abbiamo esaminato gli emendamenti che sono stati presentati dall'opposizione e ne abbiamo individuato più di uno che merita attenzione e possibilità di accoglimento. Questo, Questo, però, non significa che i lavori si debbano interrompere, perché sono proposte che man mano potranno essere prese nella debita considerazione.

non significa che bisogna fermarsi per una riflessione ulteriore. Su quei temi c'è certamente sintonia. Non è improbabile che nel corso del dibattito, da noi fortemente auspicato, possano emergere ulteriori valutazioni concordi. Chiedo all'opposizione di rendersi conto che vi è grande attenzione sul provvedimento di cui discutiamo. Non vi è ragione oggettiva per la quale si debba interrompere l'*iter* di valutazione.

vivace su un argomento complesso, che richiede un confronto - così come è stato in Commissione - anche in Aula. Non mi sembra che questo confronto denoti stanchezze di sorta, ma un interesse per una riforma che è attesa da sessant'anni. Ritengo, quindi, che oggi occorra proseguire. Il confronto sarà serrato: ben venga, questo fa parte della logica parlamentare.

l'accesso alla professione, gli esami. A tutti è noto che uno dei punti cruciali che attiene

Il tema di cui dibattiamo, su cui ci auguriamo possa trovarsi una convergenza, è quello di dare una diversa dimensione, dimensione, dignità e capacità politica al ruolo e alla funzione dell'avvocato, centrale in un processo rinnovato, che veda finalmente - questo è il nostro auspicio - una giurisdizione all'altezza dei tempi e delle esigenze del Paese. noi dobbiamo insieme, colleghi della maggioranza, trovare una via di uscita a quello che è un vero flusso inarrestabile di iscritti agli Ordini degli avvocati: 250.000 avvocati non possono essere essere del livello e della professionalità che il Paese oggi esige, anche e soprattutto per esigenze di carattere internazionale. C'è bisogno di selezionare: è prevista una formazione nuova, ma poi si prevede l'esame

docenti universitari. Io non credo che ci possa essere una terzietà, cui pure fa riferimento la norma, se lo stesso Consiglio nazionale forense è quello che deve gestire la formazione e la costituzione delle commissioni d'esame. Possiamo avere la terzietà togliendo al Consiglio nazionale forense la possibilità di nominare al suo interno sostanzialmente le commissioni. Proponiamo presso il Consiglio nazionale forense le commissioni d'esame vengano istituite a livello distrettuale dal Ministero della giustizia e siano composte, secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale, da avvocati che abbiano maturato particolare competenza ed esperienza nel settore, per il quale viene richiesto il titolo di specificazione. Questi componenti commissari vengono individuati, secondo l'emendamento 8.224, da quelli segnalati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli degli Ordini territoriali, dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari. La terzietà può essere garantita solo nella misura in cui sarà il Ministro della giustizia a gestire questa fase delicatissima della composizione delle commissioni. Ricordo a tutti i colleghi come fino ad oggi è stata regolata la questione, soprattutto fino all'ultima riforma che ha previsto - io dico: in maniera abbastanza oculata - che gli esami si tengano in un distretto diverso da quello di appartenenza dei concorrenti. fino a qualche anno fa - ma continua oggi ad esserci un aspetto molto inquietante - i commissari erano gli stessi avvocati, in prevalenza, degli stessi distretti

naturalmente, un facile accesso alla professione. Con questo emendamento crediamo di poter contribuire al superamento di tale inconveniente, di cui dobbiamo liberarci.

*(PD)*. Signora Presidente, se mi consente vorrei apporre la firma a questo emendamento e fare una dichiarazione di voto per il Gruppo del Partito Democratico. Intervengo su questo emendamento (ma avrei potuto farlo, con le stesse argomentazioni, su altre parti del provvedimento) perché siamo di fronte, anche qui, ad un tentativo di blocco all'ingresso nel settore della professione forense. Da una situazione di terzietà, neutrale, quale è quella attuale, si passa al Consiglio nazionale forense che fa l'esame e ammette alla specializzazione gli avvocati.

Il dispositivo in esame si aggiunge a una serie di altri dispositivi contenuti all'interno di questo disegno di legge - le barriere all'ingresso, le tariffe minime, il divieto alla costituzione di società di capitali - che rappresentano esattamente un insieme concettuale di limitazioni della libertà di mercato che abbiamo già sottolineato con gli ordini del giorno ma che si evidenziano palesemente in ogni passaggio del provvedimento.

molti avvocati ci fanno sapere in questi giorni che la limitazione all'apertura, per esempio, di società di capitali li pone in difficoltà competitiva con gli studi stranieri o europei.

ricadranno su tutti gli operatori economici che, non godendo di alcuna protezione, si trovano nella condizione di dover competere sui mercati internazionali avendo, però, sulle spalle i mercati monopolistici e le rendite di posizione.

di mercato, alla concorrenza, che produrrebbe una maggiore efficacia ed efficienza del sistema, e introducendo nuovi costi per la parte più debole del sistema, che è quella che compete sui mercati internazionali senza protezioni corporative,

Quindi ci troveremo persino nell'assurdo che uno studio legale italiano non può fare pubblicità nei giornali, nei mezzi di comunicazione che ciascuno ritiene più opportuni, mentre altri potrebbero farlo, per esempio degli studi legali stranieri (in particolar modo mi riferisco a studi che esistono proprio in Europa). Sul punto credo che sia utile dare un'occhiata al

come è normata in questi Paesi la pubblicità. a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale».

atipico, perché non è poi sanzionato dalla norma di legge, ma dalle sanzioni disciplinari del Consiglio nazionale forense.

In Spagna, ai sensi dell'articolo 7 del codice deontologico, l'avvocato può pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità sia dignitosa, veritiera e corretta

si può parlare soltanto più genericamente di «informazioni sull'esercizio della professione». Allora, con il comma 1 si spiega che «è consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa». Ci mancherebbe altro che un avvocato non potesse dare informazioni sule sue modalità di esercizio della professione! è davvero un paradosso: o si dice una cosa ovvia, o si vuole dire-non dire che questa informazione, in realtà, è pubblicità, però, siccome il termine «pubblicità» deve essere espunto, allora non lo si mette.

"pubblicità", che non credo sia un peccato. Non vedo assolutamente per quale motivo debba essere considerato quasi come un affronto che un legale possa pubblicizzare il proprio lavoro, il proprio studio e, in qualche modo, anche con la pubblicità dare le informazioni per raggiungere un'ipotetica ed eventuale

a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale». E poi, volendo, si potrebbe aggiungere un emendamento che interessa - stavolta davvero - non gli avvocati, ma i cittadini cittadini che si rivolgono agli avvocati. Infatti, anche il cittadino ha diritto di essere informato sulle modalità e le qualità delle prestazioni dell'avvocato e di poter comparare le tariffe anche attraverso la pubblicità.

per quello che vuol dire o far arrivare l'avvocato al suo possibile utente. Credo che questo sia il senso di una legge. Signora Presidente, la questione della pubblicità in materia di servizi legali legali è strettamente legata alla questione della specializzazione. In sostanza, si tratta di consentire che gli utenti ed i clienti possano sapere, capire sapere, capire e conoscere, anche in modo fine e puntuale, la qualità del servizio che viene offerto.

Tutta la scienza economica moderna ci dice che perché i mercati funzionino meglio e garantiscano più adeguatamente del prodotto, del bene o servizio, occorre che si favorisca una piena circolazione delle informazioni. Ora, l'articolo 9 è ispirato invece fondamentalmente a diffidenza nei confronti della circolazione delle informazioni. Già usare il termine informazioni e non pubblicità indica che si vuole sottrarre questo particolare settore di produzione e offerta di servizi al principio generale, che è quello invece della libera circolazione delle informazioni. È vero,

non attribuendo al Consiglio nazionale forense o comunque ad un organo espresso dalla categoria il compito di mettere una cappa di piombo sulla circolazione delle informazioni. Il modo

che risulta potenzialmente fuorviante e limitativo rispetto a tutto ciò che è contenuto all'interno di questo disegno di legge, in quanto non si esplicita con chiarezza la possibilità per il professionista di ricorrere allo strumento pubblicitario ai fini della promozione della propria attività,

Tutto ciò premesso, i cinque sottoscrittori dell'ordine del giorno chiedono un impegno al Governo «ad accogliere le osservazioni dell'Antitrust per quanto riguarda la disciplina della pubblicità da parte dei professionisti avvocati, e ad apportare in tal senso le opportune modifiche al testo». disegno di legge che stiamo riprendendo di settimana in settimana, anche con delle ellissi temporali che sono inspiegabili, ma che comunque avvengono, credo che abbia necessità

ripensare nottetempo ad alcuni degli articoli che possono sempre essere emendati. Questa maggioranza ce ne ha dato più volte l'esempio con dei mini o maxiemendamenti che vengono creati

che da parte degli avvocati, per l'estrema delicatezza delle funzioni a cui assolvono, vi sia un tassativo e rigoroso rispetto delle norme di carattere deontologico che presiedono all'esercizio della professione. Ripeto: tutto può essere detto relativamente alla stessa, ma certamente non può essere ridotta al rango di attività meramente commerciale o imprenditoriale. Se così è, è evidente che, nel momento in cui da un lato si chiede il più tassativo e rigoroso rispetto di norme di carattere deontologico, aventi quale primario fine la tutela della collettività, parimenti non possono che essere gli organi a cui è deputato per legge che siano rispettati quei principi di carattere deontologico i titolari del compito di indicazione di quelle forme attraverso le quali deve essere data la comunicazione da parte degli avvocati delle modalità di esercizio della professione, che devono tener conto, tra l'altro, di quegli obblighi di riservatezza che non possono che essere connessi all'esercizio della professione medesima. Questo non significa in alcun modo introdurre elementi limitativi di una concorrenza professionale che, ripeto, è concorrenza professionale e non imprenditoriale, né commerciale. Non si può, da un lato, chiedere che si rispettino principi deontologici tipici dell'esercizio delle attività libero-professionali e, dall'altro, pretendere acriticamente di imporre norme di carattere commerciale e imprenditoriale che attengono a tutt'altra materia.

Presidente, gli emendamenti 9.200 e 9.201 sono identici. Vorrei far osservare all'attenta collega Poretti, che molto si è spesa per questo emendamento, che in realtà il risultato a cui si mira è assolutamente contraddittorio. Si pretenderebbe, infatti, che la pubblicità - termine a cui tiene molto, ma non è una questione nominalistica debba essere non fuorviante (e fin qui si capisce), ma anche non incompleta. Ho un mio pensiero sul fatto della incompletezza della pubblicità:

e avanti così all'infinito. Quindi, questo criterio di incompletezza è assolutamente incomprensibile. La volete così? Vietereste la pubblicità! Volete approvare

L'emendamento 9.205, brillantemente illustrato dal professor Ichino,

sia affidato ai singoli Consigli dell'Ordine, per evitare, evidentemente, una frammentazione. Infatti, un Consiglio dell'Ordine potrebbe operare in un senso e un altro in senso completamente diverso o significativamente diverso.

Se il Consiglio distrettuale dell'Ordine è competente a controllare che l'avvocato svolga la propria attività con correttezza e lealtà in relazione a tutti gli altri aspetti del codice deontologico non si vede il motivo per cui lo stesso Consiglio dell'Ordine che, oltretutto è più vicino ai fatti, non possa e non debba essere competente per il controllo sul decoro dell'informazione della pubblicità professionale. Se il principio che regola la materia dovesse essere quello che lei ha qui enunciato,

fare soltanto una precisazione di carattere tecnico-giuridico al senatore Ichino, perché il controllo preventivo richiesto nell'emendamento

perché l'Unione europea e i principi dell'*Antitrust*, che proteggono la libertà di informazione e di pubblicità, non lo tollerano;

Tra i mali oscuri che impediscono al sistema Italia di crescere, tutti gli organismi internazionali indicano anche il difetto di concorrenza nei settori dei servizi all'impresa.

il rilievo fatto con amabile ironia dal rappresentante del Governo fosse da ricondurre esattamente in una dimensione meramente ironica nel ragionamento che si stava sviluppando. Per quanto riguarda il resto, faccio presente che una cosa è

intendo fare una dichiarazione di voto, a meno che non intenda farla anche il senatore Pistorio, se ma volesse cimentarsi a sostenere l'emendamento che ha presentato; può comunque farlo, siamo di due Gruppi diversi.

Comprendo che di pubblicità non si parli, ma è anche un po' paradossale che si preveda e si disciplini come informare. Potrebbe bastare l'articolo 21 della Costituzione per garantire il diritto all'informazione. Ovviamente, l'informazione non è pubblicità: questo tutti lo sappiamo; la pubblicità non è mera

il comma 2 dell'articolo 9, che recita: «Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza

dove si fa riferimento al cittadino, che «ha diritto ad essere informato sulle modalità e le qualità delle prestazioni dell'avvocato e a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità». Ribadisco che se voleste togliere la parola "pubblicità" sarei ben disponibile, anche perché quello che aiuta davvero l'utente a scegliere, a selezionare, ad avvicinarsi ad uno studio legale piuttosto che a un altro è sicuramente la trasparenza delle informazioni che l'avvocato dà di sé, per esempio sui siti Internet, attraverso pubblicazioni nelle riviste e nei siti di interesse giuridico

Si nega la possibilità di parlare della pubblicità, però poi, a ben guardare, quanti avvocati intervengono in trasmissioni televisive, radiofoniche, sui giornali a raccontare il loro operato

oggi, nonostante i severi moniti liberalizzatori dell'Europa, non si riesce ad accettare una figura professionale e intellettuale che si possa davvero ritenere libera di esprimersi con un proprio sito, con

Il cittadino ha diritto ad essere informato sulle modalità e sulla qualità delle prestazioni dell'avvocato nonché a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità».

non ho purtroppo la raffinatezza di linguaggio giuridico che è stata qui esibita da molti dei nostri colleghi, né sono caustico come il nostro illustre senatore Longo, però credo che vada

ad avere una legge di riforma ben fatta ed esaminata con continuità di attenzione dal Parlamento. Va contro la dignità di noi senatori, che non siamo pecore a comando, ma persone pensanti. Io credo che qui si stia giocando con la dignità di questo Senato! riprendendo un suggerimento dell'illustre senatore Longo: se vogliamo portare avanti la riforma della professione forense, forense, calendarizziamola per lunedì, martedì e anche mercoledì 2 giugno e leviamola dal calendario di questo Senato che deve affrontare la crisi economica, i rimedi per la crisi e molte altre cose fondamentali per il nostro futuro.

casi), così come le "ospitate" - per usare un brutto termine - nelle trasmissioni televisive (dai *talk show* alle trasmissioni sportive sono sempre presenti i soliti avvocati)

io credo di dover fare una riflessione: nel momento in cui è stato affermato il principio del diritto - e non solo del diritto, ma anche dell'opportunità - alla pubblicità, ritengo che poi il tutto debba essere riportato al sistema, nel senso che, stabilito che si può avendo presenti alcuni limiti di carattere deontologico (come pure è stato opportunamente ricordato), saranno poi gli addetti ai lavori, cioè l'*Authority* che di pubblicità si occupa, a regolare il sistema. onorevole relatore e rappresentante del Governo, ad un punto che è contenuto nel comma 3: la regolazione degli strumenti dell'informazione e della comunicazione. Ritengo non opportuno affidare al Consiglio nazionale forense la regolazione di questo aspetto, quantomeno, perché rischia di determinare delle conseguenze e delle soluzioni totalmente asistemiche. E questo sì, richiamando la premessa che ho fatto sulla mia confessata incompetenza alla questione, a forte rischio di violazione grave di sistemi che assicurano la concorrenza in punti centrali della nostra convivenza.

all'organo apicale dell'avvocatura, all'organo istituzionale dell'avvocatura, la regolamentazione di questo fenomeno nuovo per l'attività degli avvocati: la pubblicità. È ben vero che forme di pubblicità indiretta molto spesso recano vantaggi a soggetti che poi non ne hanno particolare bisogno (perché le prime pagine delle copertine, ove ove mai rappresentassero l'immagine di un avvocato, rappresenterebbero l'immagine di un avvocato noto e apprezzato che, appunto, si è guadagnato le prime pagine nel corso della sua carriera), la novità dello strumento impone attenzione, rigore. Impone che vi sia un organismo che dia indicazioni. Il CNF - è questa la valutazione che è stata fatta -potrà naturalmente modificare (proprio perché è depositario di questa facoltà), nel corso dei tempi che verranno, le indicazioni di opportunità che darà in un primo momento,

pubblicitarie che abbiamo avuto modo di notare nel momento in cui entrò in vigore la legge Bersani. Alcuni avvocati, ad esempio, si proponevano immaginando impegni economici molto più contenuti rispetto a risultati che sarebbero stati certamente conseguiti, ed altro ancora. È opportuno che vi sia uno strumento di controllo, un organo di controllo. Ed è per questa ragione che, pur comprendendo appieno le argomentazioni sottili, intelligenti del senatore Caruso, sono costretto a mantenere il mio parere contrario. comprendo l'esigenza manifestata dal senatore Caruso. Vorrei però ricordare a me stessa

abbiamo fatto in base ad un ragionamento. Ci siamo cioè posti il problema di come la pubblicità o l'informazione possa essere attuata dai vari avvocati, e ci siamo chiesti se era possibile che un Consiglio dell'Ordine ritenesse lecito un determinato comportamento secondo un'interpretazione del codice del codice deontologico e un altro Consiglio dell'Ordine, magari di una città diversa, lo ritenesse invece illecito, sempre in base ad una interpretazione del codice deontologico. Proprio per uniformare,

Senatore Caruso,

Non facciamo pasticci. Prendiamoci il tempo necessario e voteremo nella prossima sessione dedicata a questo

per dire che nel pur lento, ma importante, progredire dell'esame di questa rilevante legge, non è tempo perduto sottolineare e solennizzare in qualche modo la conclusione dell'esame dell'articolo 9. È molto importante ed è molto emblematico, in quanto raccoglie discussioni di anni, più che di mesi, e si arriva ad una conclusione assai significativa. Naturalmente non può essere soppresso il comma 4, che è quello che prevede la sanzione («L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare»), altrimenti le precedenti statuizioni non avrebbero sanzione e non avrebbero vigenza ed efficacia. Ma in questo articolo 9 finalmente si stabilisce prima di tutto, e non è questione terminologica, che non è dato fare pubblicità. È molto importante che questo concetto rimanga estraneo al mondo dell'informazione riguardo alla professione forense. Si stabilisce, sono le prime due parole del comma 1 dell'articolo, che «È consentito» - è dunque una facoltà - esercitare questa possibilità di informazione, ma non già si stabilisce un obbligo al quale sarebbe correlato un diritto degli interlocutori, di coloro che forniscono la prestazione forense. Il principio fondamentale di questa di questa legge e di questo articolo è il seguente: si intende che l'avvocato, che il professionista, nella sua consistenza, nella sua dignità, nella sua figura, nella sua rispettabilità acquisisca clientela in virtù di una qualità che si afferma, si dimostra, si propaga, anche si comunica, ma non in virtù di una pubblicità promozionale. È coerente da parte di coloro che hanno una visione commercialistica della professione, di una falsa liberalizzazione introdotta nella materia, sostenere la volontà di fare *promotion*, di acquisire clientela non tanto per il buon nome o per la dignità o la comprovata capacità o qualità del professionista, ma per lo sforzo pubblicitario. Sono gli stessi che andavano sostenendo le società di capitali e gli investimenti economici a questo riguardo, come regola fondamentale. Infatti, una società di capitali ben può investire grandemente sulla pubblicità per l'appunto, a prescindere dalla qualità, dalla dignità e dall'attendibilità professionale del professionista o dei professionisti che dovrebbero essere promossi. Lo riconosco, senatore Ichino e altri, che vi è una coerenza nel vostro atteggiamento, ma è giustamente contraria al principio informatore di questa legge.

che vedono riportata la propria immagine o le proprie parole sui grandi mezzi di informazione. Lo so, questo sì, questo è vero, ma non riguarda solo la professione forense. che dire del mondo della politica, in cui 15 persone sono tutte le sere sui telegiornali e le altre navigano nella onorata sconosciutezza? E così in tanti altri settori della vita pubblica, BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. ...o l'altro settore, ma di questo non dobbiamo fare carico al ceto forense o ad altro ceto professionale. Semmai ne dobbiamo far carico ai mezzi d'informazione, al sistema della comunicazione pubblica e dell'informazione, che rivendica sempre la propria libertà, ma in realtà va soggetto a regole tutt'altro che deontologiche nel disciplinare la propria attività. L'articolo 9 è pertanto molto importante e rappresenta una tappa significativa nella riforma dell'ordinamento forense

i criteri e le modalità di applicazione. È importante che respingiamo l'emendamento 9.213, ma soprattutto che approviamo l'articolo 9 nella sua interezza.

la concezione commercialistica o non commercialistica della professione, ma soltanto il fatto che voi avete la pretesa che si possa garantire per decreto la qualità della professione forense, mentre noi siamo convinti che in tutta la storia dell'economia in tutta la storia dell'economia su questo pianeta non si sia mai trovato altro sistema per garantire la qualità delle prestazioni, dei servizi, di ciò viene offerto e acquistato, se non la libertà di circolazione delle informazioni in proposito. Voi state limitando la libertà dell'informazione e, di conseguenza, la possibilità di miglioramento e di controllo sulla qualità delle prestazioni forensi.

il senatore Segretario sta ritirando delle schede.

Colleghi, per cortesia.

Signora Presidente, non ho le capacità di tattica parlamentare della collega e quindi, da banale lavoratore di questo Senato, illustro gli emendamenti che ho scritto e proposto all'attenzione dei

dedicato a decine di migliaia di avvocati che, con onestà e dedizione, quotidianamente svolgono il proprio lavoro, per sé, per le proprie famiglie

L'articolo 10 si dedica alla formazione permanente, che è un argomento che, in generale, occupa i

alla formazione permanente gli avvocati iscritti negli albi speciali per il patrocinio davanti alla suprema Corte di cassazione. Non ve ne è una ragione apprezzabile credo che il praticare la professione davanti alla suprema Corte imponga una formazione specialistica e particolare e forse, in alcuni casi, superiore a quella generalista richiesta ad ogni avvocato. Gli emendamenti 10.221 e 10.224 propongono al relatore, al Governo e ai colleghi di rimuovere un'aporia che mi sembra essere contenuta nel testo, la norma propone che siano esentati dagli obblighi di formazione i consiglieri regionali, e non già gli assessori regionali. Se il metro per l'esonero è quello dell'impegno che l'amministratore pubblico profonde in tale versante della sua attività, credo che sia indubitabile che quella degli assessori regionali sia un'attività di gran lunga assorbente.

attività, un *new business* che si è affacciato anche e soprattutto all'interno delle nostre professioni. Credo che i Consigli degli Ordini e coloro

è un luogo privilegiato di formazione che mi sembra non possa essere escluso dall'alveo di attenzione di questo provvedimento.

Saccomanno, rimandando alle osservazioni fatte in sede di discussione sulle specializzazioni. Credo che con «altri soggetti» possa evidentemente intendersi anche l'università

Non sono contrario a questa specificazione. Si tratta di un argomento che avrei voluto trattare quando è stato affacciato con riferimento alla formazione specialistica. Sono assolutamente d'accordo, non contrario, al fatto che l'università sia coinvolta in questo contesto, anzi direi che sono favorevole, mi sembra una cosa logica. Credo che, però, ogni cosa debba essere collocata al suo posto. Ricordo ai colleghi

occupa specificamente di questo, cioè delle relazioni tra il Consiglio nazionale forense, gli Ordini e le facoltà di giurisprudenza. Ritengo che quella sia la sede propria per inserire una disposizione di questo tipo, affinché la legge che risulterà dai nostri lavori abbia buoni e opportuni vocaboli e armonie interne. Credo che gli avvocati e la professione forense meritino anche questo: una buona qualità di formazione di formazione legislativa.

il Ministero della salute riconosce diritti per complicanze irreversibili derivate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati. Questi cittadini hanno deciso di accedere alla transazione di cui alla legge n. 244 del 2007 e aspettano che siano riconosciuti i loro diritti

ma, detto questo, scende poi il silenzio più drammatico degli uffici. Questi cittadini oscillano tra i loro legali e inutili telefonate al Ministero. Finalmente, magari dopo vent'anni, gravemente ammalati, viene loro riconosciuto un diritto e, beffa nel riconoscimento del diritto, non accade nulla. Ho citato il caso della signora Bertone di Mondovì, ma da moltissime parti in Italia ci giungono le stesse segnalazioni. Seguirà un'interrogazione, e speriamo che questo possa sveltire la grigia

Formica, è stato finalmente assolto dopo 17 anni di processo. Sedeva nel nostro Parlamento, come siede nel nostro Parlamento la persona a cui si devono le iniziative giudiziarie che hanno portato ad una assoluzione per non aver commesso il fatto. Non è il solo caso di gravissima malagiustizia che ha toccato la politica italiana: 17 anni atteso per essere assolto Rino Formica, 17 anni ha atteso per essere assolto Calogero Mannino.

sì, la soddisfazione di essere stato assolto, ma sono stati 17 anni di gogna. Il suo non è stato un caso personale, ma

per malagiustizia. Tutte le accuse contro Rino Formica si sono rivelate inconsistenti. Qui, in quest'Aula, siede la persona che ha portato avanti quelle accuse. E mi domando se quella persona oggi senta la necessità non dico di pentimento, ma almeno di turbamento per aver distrutto la personalità di Rino Formica e per averlo tenuto fuori dalla politica, che era la sua vita, per 17 anni.